L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

sociale. Esso è volto ad evitare che questa fondazione sia alimentata anche da risorse pubbliche, a parte la dotazione iniziale di un milione di euro. Non si tratta di essere contrari al fatto che vi possano essere *partnership* tra pubblico e privato, ma all'idea che risorse pubbliche siano gestite da soggetti terzi, anche e specialmente quando vanno a favore del terzo settore. Il modo in cui il settore pubblico eroga risorse al terzo settore avviene attraverso procedure di evidenza pubblica e di bandi trasparenti e non si affida alla discrezionalità di un soggetto terzo.

Saluto i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Gabriele Faggella» di San Fele, in provincia di Potenza, che stanno assistendo ai nostri lavori.

nell'ambito di quel centrosinistra che dovrebbe esprimere questa maggioranza di Governo, ma molto a destra; uno si dice organo del del socialismo nazionale; ma dal contesto sembra più del nazionalsocialismo che del socialismo nazionale e non so se anche questo piace. Tuttavia, al di là dei nomi,

ridurre ulteriormente i pochi strumenti di controllo e di verifica per il Parlamento e per il Paese nei confronti dell'attività di questa fantomatica fondazione.

dell'altrettanto fantomatico organismo dirigente di questa fondazione. Insomma, una vera porcheria, buttata lì, nell'ambito di un provvedimento già piuttosto confuso, con una delega in bianco al Governo, totalmente estranea a quel che dovrebbe approvare un Parlamento. Presidente, non ripeterò le considerazioni poc'anzi esposte dal senatore senatore Malan, che in buona parte condivido. Cercherò di non annoiarvi e di dire soltanto ciò che ritengo necessario e, modestamente, originale. Qui si istituisce per legge una fondazione che ha le caratteristiche di un ente privato che tuttavia riceverà finanziamenti pubblici e già questo mi sorprende. Ma come ente privato, essa potrà procedere ad assunzioni senza bando ed avrà tutta la libertà, l'autonomia

Mi chiedo chi sarà il presidente di questa fondazione, chi comporrà il consiglio di amministrazione. Qualcuno già dice che ci sarà quel Vincenzo Manes che - se non ricordo male - con oltre 60.000 euro ha finanziato la fondazione politica del Presidente del Consiglio. E se non sarà lui saranno altri dell'*entourage* fedeli alla Leopolda. Me lo suggerisce anche un altro fatto: con un curioso *lapsus* si dice che lo statuto della Fondazione sarà approvato «con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri del lavoro e delle politiche sodali». «Sodali»! Signori, qui stiamo parlando di un crogiuolo clientelare, che nulla ha a che vedere con le virtù del terzo settore. Stiamo parlando di uno strumento elettorale, uno strumento per muovere capitali. Da questo testo non capisco che cosa impedirà a questa fondazione di finanziare, ad esempio, i progetti

impatto sociale e occupazionale conseguito, ma sarà facile dimostrare e opinare, perché non c'è nulla: questa non è nemmeno una delega, è una norma ed è così vaga ed inconsistente che pensar male non soltanto è possibile, diventa quasi un dovere prudenziale.

esaminando un disegno di legge e non una legge delega, che diventa, alla fine, semplicemente un cavallo di Troia per veicolare interessi politici di parte. Ho sentito tanti colleghi indignarsi per questo e promettere battaglia, ma non vedo il calor bianco che mi sarei aspettato e me ne

In primo luogo consideriamo l'istituzione della Fondazione Italia sociale del tutto estranea all'oggetto del disegno di legge in esame, che riguarda il terzo settore. È chiaro che nessuno avrebbe potuto vietare al Governo di istituire l'ennesima fondazione pubblica, con lo scopo di raccogliere fondi, soprattutto tra i colossi della finanza, ma questa è un'operazione differente dal terzo settore e dalla discussione svolta in questi giorni. L'una è un'operazione di solidarietà filantropica, l'altra è un'operazione un'operazione di solidarietà, caratterizzata dalla partecipazione attiva dei cittadini. Lo abbiamo detto in tutte le nostre discussioni: se c'è un elemento che caratterizza oggi il terzo settore e quindi lo distingue anche da altre forme particolari - da ciò deriva anche la nostra

pone anche un problema di merito, che vogliamo sottolineare ancora una volta. Se questa era l'idea principale del Governo e della Presidenza del Consiglio, che ha anche un incarico specifico

Signor Presidente, qui sorge proprio il dubbio se venga prima l'uovo o la gallina. Sembra quasi che questa legge delega sia stata fatta su misura per calarvi all'interno un emendamento di questo tipo. Un emendamento che abbiamo considerato subito, già nella prima versione che poi è stata ritirata in Commissione, come irragionevole e non avente nulla a che fare con gli obiettivi prefissati dal disegno di legge in esame. Con questo emendamento si interviene per istituire l'ennesimo carrozzone, finanziato sempre con i soldi pubblici dei contribuenti, senza che siano definiti in modo chiaro ed esplicito compiti e funzioni. Con questo emendamento si delega a un decreto ministeriale l'approvazione dello statuto della Fondazione, senza fissare principi e criteri direttivi puntuali si prevede inoltre lo stanziamento di un milione di euro per la dotazione iniziale per l'anno 2016, cifra non da poco. La libertà di agire come vuole di chi guiderà questo carrozzone è sicuramente impressionante. La parola d'ordine sarà sicuramente: appalti. Noi siamo ovviamente contrari, come abbiamo già sostenuto in Commissione. È un emendamento che non trova ragione di esistere in una legge come questa.

Signor Presidente, secondo i più recenti dati disponibili, in Italia operano oltre 6 milioni di volontari e 300.000 enti del terzo settore. I centri di servizio per il volontariato sono 74 (72 quelli aderenti al coordinamento nazionale) e nel 2013 hanno offerto servizi a 43.000 organizzazioni e 23.364 cittadini, promosso 5.576 interventi a favore del volontariato e coinvolto ben 154.492 studenti. Hanno erogato, inoltre, 29.708 ore di formazione e 12.981 servizi servizi di orientamento e consulenza. A loro oggi questo disegno di legge deve dare risposte e avrebbe dovuto darne sicuramente di più di quelle che, fino a questo momento, con gli emendamenti approvati, sono state fornite. Noi crediamo che le aspettative di quanti operano nel mondo del volontariato in relazione ad una riforma del terzo settore, richiesta da tempo anche in virtù di mutate esigenze sociali, siano state ampiamente disattese. Nonostante le modifiche apportate alla Camera, il testo risulta ancora ampiamente deficitario dei principi e criteri direttivi necessari per una corretta, univoca e non arbitraria identificazione degli enti del terzo settore, che ne tracci con chiarezza la distinzione rispetto alle imprese e agli enti con finalità lucrative nel rispetto dei principi di certezza del diritto e di leale concorrenza. Questo, affinché agevolazioni e sgravi tributari siano assicurati solo alle organizzazioni che perseguono esclusivamente finalità di promozione del bene collettivo, elevazione dei livelli di cittadinanza attiva, coesione e protezione sociale. Ma tanto più non è proponibile oggi che il disegno di legge delega viene presentato a quest'Assemblea con la sorpresa finale, quella che ha destato le preoccupazioni delle ultime ore, ossia l'introduzione, attraverso l'emendamento, della Fondazione Italia sociale che pur è stata corretta, rispetto all'iniziale previsione, con gli emendamenti discussi fino a qualche minuto fa. L'ottimo relatore Lepri ha cercato di attutire e ridimensionare la portata di quell'emendamento e di migliorare complessivamente il disegno di legge; ciò nonostante restano diversi rilievi negativi, attinenti sia sia il merito della riforma. Nel metodo non si può non rilevare che il confronto con il variegato e molteplice mondo del terzo settore è stato certamente compresso nei tempi e nella qualità dell'interlocuzione e non si è tenuto debito conto di tutte le proposte e i suggerimenti provenienti dai veri attori del settore, cui, poi, questa riforma è realmente dedicata. Il disegno di legge evidenzia particolari difetti anche nel merito delle scelte operate dal Governo e rifinite nel precedente passaggio alla Camera. quest'Assemblea rischia di perdere ancora un'occasione preziosa per fornire risposte più precise e concrete alle migliaia di volontari che si attendono di vedere riconosciuti e sostenuti i principi e i valori che ispirano il loro lavoro. Eppure, proprio dal Forum nazionale del terzo settore è arrivata forte la richiesta di una riforma condivisa con i suoi destinatari (per questo parlavo prima di problemi di metodo che riguardavano un maggior confronto).

seppur modificata con i subemendamenti. certamente la scelta di istituire per legge una fondazione, attraverso anche una *start-up*, poteva creare una fase di disorientamento, e così è stato nel corso della discussione, prima in Commissione e poi in Aula. Sono nate in tal modo diverse perplessità. I rischi di questa operazione potevano essere uno il contrario dell'altro: il primo, pensare che la fondazione potesse attrarre un flusso considerevole di donazioni private, anche perché

Altre ancora possono essere le criticità della riforma da evidenziare in questo ultimo scorcio di dibattito. Nel disegno di legge non si fa alcun cenno ad una previsione di semplificazione della procedura di acquisizione dello *status* di organizzazione non governativa, come pure ad una revisione del sistema di gestione dei beni confiscati alla mafia, in quanto si ritiene che il Governo debba adottare una maggiore razionalizzazione della gestione degli stessi beni. Uno dei maggiori problemi resta quello di consentire anche ad associazioni di nuova costituzione e gestite da giovani la possibilità di accedere all'acquisizione del bene per poter avviare un'attività *no profit*. Si continua a creare forte confusione tra la stabile e prevalente attività di impresa e le attività tese al solo autofinanziamento delle associazioni, che rappresentano la vera forma di autosostentamento Viene attribuito anche scarso rilievo al profilo partecipativo che, invece - come sostengono giustamente le associazioni di volontariato -, è il motore dell'attivazione dei cittadini e un prerequisito per tutto il terzo settore. Il disegno di legge, inoltre, differenzia lo *status* di volontario non in base alle attività svolte, bensì in relazione alla tipologia di organizzazione in cui opera, rischiando in tal modo di creare una differenza tra volontari di serie A e volontari di serie B. L'introduzione del Consiglio nazionale del terzo settore può rappresentare una positiva innovazione come luogo di incontro e di raccordo con le istituzioni, ma non deve categoricamente sovrapporsi agli organismi di rappresentanza del terzo settore. Non ci convincono, peraltro, le parti che riguardano la distribuzione degli utili, il tema della sussidiarietà attraverso il coinvolgimento di cittadini, imprese, investitori e operatori del settore *no profit* e una diversa partecipazione alla fiscalità. Anche qui ci sarebbe da dire molto di più. Noi riteniamo che si debba procedere ad una revisione completa attraverso una verifica puntuale di tutti gli enti/associazioni iscritti all'albo del 5 per mille. Sono migliaia le associazioni iscritte a questo registro, gestito dall'Agenzia delle entrate, che ottengono, come sappiamo, proventi derivanti dal cinque per mille senza effettivamente provare il reimpiego di questi proventi per utilità sociale (si aprirebbe tutta una discussione sull'effettiva utilità del gettito del 5 per mille). Inoltre, occorrerebbe rendere più efficiente l'erogazione dei fondi, comunque sempre esigui. Le finalità indicate nel disegno di legge delega erano tutte condivisibili nel complesso; abbiamo detto, infatti, in diversi interventi, che auspicavamo una riforma del terzo settore e che condividevamo la *ratio* originaria sulla necessità di riforma dello stesso. Tuttavia, molte di queste aspettative sono state tradite. Questa riforma doveva servire a fare chiarezza e a riorganizzare compiutamente i centri servizio la cui funzione solidaristica viene modificata e addirittura in alcuni casi stravolta, creando una confusione di ruoli. Doveva servire a semplificare, sostenere e favorire il volontariato, proteggendolo dagli abusi, dalle cattive prassi

la condivisione della necessità della riforma, riaffermiamo comunque i rilievi negativi fin qui illustrati e prendiamo atto che c'è stato *in limine mortis*, con gli ultimi emendamenti, qualche segno di attenzione, attenzione, anche per un subemendamento del nostro Gruppo. Ma nel complesso, avendo data ampia espressione di non condivisione rispetto a tutti gli articoli del disegno di legge, non possiamo che confermare il nostro voto complessivamente contrario, pur apprezzando gli sforzi

Signora Presidente, colleghi, è già una sorpresa che su questo provvedimento non sia stata messa la fiducia. Come abbiamo avuto modo di spiegare nell'illustrazione delle nostre pregiudiziali, il il disegno di legge del quale concludiamo l'esame presentava diversi profili di incostituzionalità, come abbiamo ribadito più volte. «L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti»; così recita testualmente Ma anche questo è andato in cavalleria. In ragione della complessità della materia trattata dalla delega, i principi e i criteri direttivi alla base di tale provvedimento ci sono apparsi e ci appaiono ancora talmente ampi e generalistici da far presupporre l'impossibilità effettiva di rispettare la legge di delegazione, producendo nei fatti un eccesso di delega che, se sottoposta al giudizio della Corte costituzionale, chiaramente con occhi di un certo tipo, ne comporterebbe sicuramente ed inevitabilmente una dichiarazione di illegittimità. Il presente disegno di legge prevede soluzioni inadeguate, come quella di accentrare le competenze a livello statale, istituendo un registro unico ed affidando all'Agenzia delle entrate e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il controllo sull'andamento delle attività, senza del resto istituire nessun organo specifico di vigilanza. Esso contiene inoltre interventi disomogenei rispetto al contesto della riforma, che prevede la trasformazione del servizio civile in servizio

Le disposizioni nell'ambito del servizio civile ci appaiono sganciate dal contesto del disegno di legge delega e non organiche. indicati i criteri e i principi direttivi generali non si fa alcun riferimento al tema della revisione del servizio civile, né vengono citati gli articoli 52 e 11 della Costituzione, che rappresentano la struttura portante dell'istituto. Se il Governo poi ipotizza di esercitare questa delega in bianco per normare magari la partecipazione di extracomunitari a questa comunità, esso viola secondo noi palesemente il rispetto della sovranità nazionale e il concetto stesso di identità che devono invece caratterizzare un istituto come quello del servizio civile, nato dalla volontà di istituire un sistema alternativo alla leva obbligatoria. La previsione di un registro unico del terzo settore, al fine di favorirne la piena conoscibilità in tutto il territorio nazionale, oltre ad apparire in contrasto con il rispetto delle prerogative delle Regioni, ai sensi anche della disciplina costituzionale prevista dal Titolo V, non definisce la natura giuridica dell'iscrizione e quale sia l'ambito soggettivo degli enti obbligati alla registrazione. Ci saremmo aspettati, signor Presidente, una riforma in grado, da un lato, di restituire al terzo settore la dignità della sua missione, volta, nel rispetto del principio della sussidiarietà orizzontale, ad assorbire il *gap* di intervento statale sulle questioni di impatto sociale e, dall'altro lato, di garantire formule di controllo e vigilanza sulla degenerazione che nel tempo hanno investito il mondo del *no profit*. Per quanto riguarda il servizio civile, siamo ancora più perplessi. Forse non tutti sanno che da almeno sette anni oltre il 90 per cento degli enti di servizio civile sono monitorati, gestiti e controllati non dallo Stato centrale bensì dalle Regioni. Stiamo parlando della totalità degli enti locali, perché il servizio civile, checché ne dicano molti cosiddetti esperti, è svolto almeno nel 50 per cento dei casi presso gli enti locali e dalla miriade di organizzazioni *no profit* a dimensione regionale e subregionale.

Il controllo lo si fa stando sul territorio, operando su di esso, e in questo le Regioni rappresentano sicuramente lo strumento migliore e più adatto; altrimenti accadrà quanto già accaduto in passato, ossia uno spreco di risorse pubbliche. Nel recente passato sono state decine le interrogazioni parlamentari che hanno denunciato abusi, sprechi ed omissioni nel piccolo mondo del servizio civile, quasi sempre ad opera di realtà che teoricamente dovevano essere controllate da qualche soggetto seduto a qualche scrivania dei palazzi romani. Mantenere l'attuale quadro di delega alle Regioni fa bene allo Stato, ai territori della nostra comunità, ma soprattutto fa bene ai nostri ragazzi, ma tutto ci siamo stracciati le vesti per indicarlo in parecchi emendamenti, non è stato

Questo sarà il *leitmotiv* che porterà questa legge ad essere revisionata molto presto. Il *no profit* è diventato nel tempo una colonna portante nel nostro Paese: 4 milioni di volontari e 10 milioni di lavoratori (incluso l'indotto) un proficuo esempio di tutela della cultura e dei servizi sociali. Una riforma era necessaria: questo ce lo siamo detti già da qualche anno,

Ma la legge delega che il Governo sta imponendo al Parlamento di riforma ha solo il nome, perché pare che in alcuni passaggi il *no profit* venga trasformato in *profit*. il punto di arrivo sia sempre la parola «appalti», come ho ricordato prima; per non parlare della conseguenza sleale che alcune cooperative e ONLUS potrebbero fare nei confronti di altre aziende godendo di fiscalità agevolata; l'avrete notato negli emendamento che abbiamo presentato. Ne abbiamo presentati parecchi anche sul tema del servizio sociale aperto alla questione immigrati, che probabilmente

la pausa pasquale abbia fatto passare in secondo piano le difficoltà che il Governo e la maggioranza hanno avuto in Assemblea la settimana scorsa. Il sottosegretario Pizzetti ha chiesto e ottenuto dall'Assemblea l'accantonamento dell'articolo 6 e, di conseguenza, il voto sull'articolo 7. Il Governo è stato apostrofato come pasticcione. Il provvedimento provvedimento passerà alla storia di questa Aula per l'ingresso ufficiale in maggioranza di un altro Gruppo, non senza polemiche. Questa sì che è un'opera solidaristica e sociale. terzo sistema, *no profit*, senza scopo di lucro, non governativo e non imprenditoriale sono alcune delle espressioni e dei modi per identificare tutta questa realtà che, all'interno del nostro sistema socioeconomico, si colloca a metà Stato e Regioni. Noi ci siamo posti anche un altro problema:

ci siamo chiesti, parallelamente a questo: dove sono un piano industriale, sull'energia, una strategia per l'Europa? Nulla di tutto ciò sperato che questa legge fosse buona. Avrebbe potuto rilanciare un terzo settore che è di importanza vitale e a cui troppe volte si demandano

per tantissime persone dello stare in una società complessa, articolata e soprattutto frizzante sotto tutti gli aspetti.

alle fondazioni francesi. Non facciamo inutili paragoni: la Francia è un'altra questione, un'altra storia, un altro sistema e ha un altro volontariato. Secondo il nostro Gruppo, questo non è assolutamente un paragone da fare. visto, purtroppo nella nostra triste realtà, come dietro alla collaborazione e al voler aiutare gli altri, ci sia semplicemente un voler approfittare e guadagnare sulle spalle di parecchi soggetti. Ci fa anche specie che questa questione non sia stata presa

il terzo settore è diventato sempre più centrale nell'economia e nella società italiana negli ultimi venti anni. Oggi al *no profit* si assegnano compiti essenziali sul lavoro, la sanità, l'*housing* e la cultura. Con una spesa pubblica decrescente e con uno Stato ipertrofico ma inefficiente, l'assolvimento di questi compiti diventa per molti aspetti cruciale. L'obiettivo di questa riforma è ambizioso, perché prevede di costruire un nuovo modello di *welfare* partecipativo, fondato su una *governance* sociale allargata per valorizzare il potenziale di crescita e occupazione proprio dell'economia sociale e delle attività svolte dal terzo settore che, non a caso, è l'unico comparto che negli anni della crisi è riuscito a crescere. Dunque, un serio riordino delle regole che lo disciplinano può creare nuove opportunità di lavoro, facendo finalmente decollare l'impresa sociale.

Tutti questi provvedimenti andavano nella giusta direzione, perché rimettevano in mano alle associazioni del terzo settore e alle imprese sociali la possibilità di essere protagoniste del loro destino e collocavano a pieno titolo le imprese sociali all'interno del terzo settore. Credo sia però utile chiedersi perché una così buona legge ha prodotto meno effetti positivi di quanto si poteva sperare. Il primo motivo va ricercato nell'impossibilità di distribuire utili.

inoltre dimostrato erroneo impedire ogni forma di agevolazione dal punto di vista dell'IVA e di altri vantaggi che il regime ONLUS consente e che, invece, le imprese sociali non possono adottare. questa riforma, togliendo tali vincoli, dà finalmente piena cittadinanza al concetto di impresa sociale nel terzo settore, introducendo la possibilità anche per le società a responsabilità limitata o società per azioni di remunerare il capitale esattamente nel limite previsto per le cooperative a mutualità prevalente,

Il fatto che chi mette soldi possa ricevere dividendi calibrati alla dimensione e alla realtà di un settore, insieme così atipico e così centrale, può rappresentare un elemento in grado di orientare il flusso di investimenti verso il *no profit* anche il tentativo di andare nella direzione di un uso responsabile del denaro da parte dei cittadini, delle imprese e degli investitori che devono essere aiutati con meccanismi di incentivo fiscale. Il lungo e articolato dibattito che si è svolto in Assemblea sull'articolo 6 è stato dunque in alcune parti surreale, perché l'impresa sociale fu inclusa nel terzo settore già dieci anni fa da un Governo di centrodestra. Ebbene, qui si valorizza la realtà del terzo settore consentendogli di mutuare forme organizzative tipiche delle aziende. È innegabile che finora il mondo del *no profit* abbia visto spesso le buone intenzioni fare premio sulla necessità dell'efficienza ed è altrettanto innegabile che i vantaggi, anche di tipo fiscale, molto spesso abbiano condotto a casi ambigui, nei quali *no profit* era la forma, ma non la sostanza. C'è il rischio che con la nuova normativa queste ambiguità divengano strutturali? A noi sembra il contrario, e cioè che il provvedimento in esame faccia finalmente chiarezza, anche perché il vincolo è per tutti quello della mutualità prevalente, consentendo così di eliminare sovrapprofitti che avrebbero snaturato la vocazione del terzo settore. I concetti veri su cui dobbiamo basarci per valutare il provvedimento in esame sono quindi essenzialmente due: la misurabilità dell'efficacia delle azioni poste in essere dalle associazioni del terzo settore e il dato della trasparenza. Da questo punto di vista, forse questa è un'occasione mancata, in quanto sembra essere giunta l'ora di tagliare antichi cordoni ombelicali e vecchi collateralismi politici con una parte del mondo delle cooperative che ha lucrato vantaggi spesso male usati, che hanno finito per danneggiare l'intero mondo del terzo settore.

Un altro punto critico è l'assenza della figura di un'autorità garante del terzo settore che abbia ampi poteri di controllo e garanzia su enti, procedure di affidamento e spese. Le funzioni di controllo e monitoraggio vengono assegnate

il servizio civile universale. Infine, il Governo ha presentato in 1a Commissione e poi in Assemblea un emendamento che di fatto istituisce l'IRI del terzo settore con la Fondazione Italia sociale. Si tratta di una vera e propria IRI del terzo settore, una sorta di filtro tra chi in Italia si occupa di sociale e chi lo vuole finanziare. Una materia di natura privatistica che diviene regia pubblica non può che suscitare dubbi e l'emendamento del Governo mostra un'impostazione fortemente accentratrice, una chiara tendenza al dirigismo. Rispetto al testo presentato in Commissione sono scomparsi gli apporti dello Stato, ma i soggetti pubblici sono rimasti e questo è in contraddizione con quanto sostenuto dal relatore, il quale aveva detto che, se si intende incentivare la donazione da parte di privati, imprese e cittadini, sarebbe irragionevole consentire la destinazione di risorse anche da parte di soggetti pubblici. Su questo punto, dunque, i margini di ambiguità restano molti ed è assolutamente indispensabile che il decreto con cui si darà vita alla fondazione passi dal Parlamento e sia prevista una valutazione oggettiva dell'impatto sociale delle sue iniziative. Tuttavia nel

colleghi senatori, consentitemi di introdurre questa dichiarazione di voto riferendomi a un aneddoto di tipo familiare. Durante queste vacanze di Pasqua la mia seconda figlia di diciassette anni mi ha detto

ha un connotato sociale, anche il laboratorio di una *start-up* di giovani studenti, così come una grande multinazionale. Chiunque dia lavoro, produca beni o servizi per i cittadini, chiunque si sforzi ogni giorno di stare al passo con una concorrenza sempre più agguerrita in un mondo sempre più globalizzato, chiunque cerchi di emergere puntando all'eccellenza svolge un ruolo sociale, perché contribuisce allo sviluppo del territorio e di una comunità, sia questa intesa come il suo vicinato, sia intesa come mercato internazionale. Dunque ogni impresa economica ha una funzione sociale, perché il profitto non è lo sterco del diavolo e perché chi intraprende, se lo fa secondo le regole e la legge, dà occupazione e consente la circolazione delle risorse. Ciò detto, cos'è una legge che tutela l'impresa sociale? Nel 2006, con questa etichetta di impresa sociale si era inteso una sorta di riconoscimento di merito a quelle imprese che, con qualsivoglia *status* giuridico, operavano in determinati settori considerati di utilità sociale e per questo avrebbero potuto avvalersi anche di lavoro volontario, coinvolgendo persone disabili e rinunciando alla tradizionale spartizione degli utili

chiaramente il senatore Luigi Marino quando ha sostenuto che l'impresa sociale nel nostro Paese è stata sostanzialmente un fallimento a causa della sua natura ambigua e bipolare. Dunque, cosa avremmo dovuto fare noi legislatori in questa occasione? Io credo che noi avremmo dovuto ancor più porre un discrimine garantendo che l'impresa sociale effettivamente sia quella senza finalità di lucro. Avremmo dovuto, cioè, comprimere fino a tentare di annullare quella sorta di zona grigia

avrebbe consentito di salvaguardare nella sua vera dimensione e nella sua vera essenza il volontariato, che è parte integrante del nostro tessuto culturale e delle nostre tradizioni, ed è anzi un patrimonio - lo possiamo dire oggi, nel cuore di una lunga crisi che è durata ormai più delle guerre mondiali dello scorso secolo secolo - senza il quale il nostro Paese avrebbe faticato a reggersi, e la cui importanza è diventata ancor maggiore nel difficile frangente che abbiamo In tempi di crisi economica e di sempre minore disponibilità di fondi pubblici, il terzo settore ha svolto e svolge un ruolo complementare, se non addirittura suppletivo, nel fornire ai cittadini *welfare* e servizi indispensabili, soprattutto per ciò che concerne gli strati più deboli Il *no profit*, insomma, è il luogo in cui meglio prende corpo il principio di sussidiarietà orizzontale tutelato dall'articolo 118 della nostra Carta

disegno di legge sia andato in direzione assolutamente opposta. Anziché valorizzare il volontariato nella sua essenza, anziché partire dal fatto che l'elemento distintivo della economia sociale è la mancanza di profitto ed il reinvestimento di tutti gli utili, siamo andati oggettivamente ad allargare quella zona grigia e l'abbiamo fatto prevalentemente rinunziando alle nostre prerogative di legislatori. L'abbiamo fatto quando abbiamo pensato di poter risolvere il problema dando una delega al Governo, ancor peggio una delega volutamente generica, confusa,

prive di scopo di lucro. Al contrario, nella delega abbiamo detto che è consentita una redistribuzione degli utili, magari per garantire qualche posto all'interno di queste strutture. noi crediamo di poterci salvare l'anima dicendo che gli amministratori devono rispettare il vincolo di destinare gli utili prevalentemente sottolineo «prevalentemente» - al raggiungimento di obiettivi sociali? Siamo ingenui se pensiamo che i cittadini non si rendano conto di cosa si celi dietro espressioni così generiche e così volutamente ambigue. Ed oltre che ingenui, siamo anche ipocriti, perché in questo modo stiamo offendendo sia chi fa sana impresa, sia chi svolge volontariato vero. Non solo: secondo alcune proposte contenute nell'articolo 7, si vorrebbero escludere escludere anche le imprese con finti scopi sociali dalle normali attività ispettive, cui i nostri imprenditori sono ogni giorno sottoposti. Signora Presidente, di fronte a questo passa persino in secondo piano quel servizio civile universale, istituito dall'articolo 8 del disegno per servire la nazione non in armi e poi magari averne un vantaggio in un concorso per entrare all'interno di una cooperativa o di una ONLUS. davvero, la demagogia rischia di sfociare nel ridicolo, perché, signor Presidente, la resistenza non in armi, nella storia, è stata fatta da cittadini inermi, che si sono battuti

che segna ancor di più e ancora una volta il cedimento anche culturale dell'Occidente, di fronte ai conflitti che veramente viviamo in questo secolo. Il servizio civile non in armi è stato fatto da quell'archeologo perso la vita per salvare la nostra civiltà. *(Applausi)*. Il servizio civile non in armi è stato fatto da quanti non cedono alla demagogia di un pacifismo di bassa lega,

cari colleghi, che questa legge renderà ancor più difficile per i nostri cittadini alzarsi ogni mattina per andare a sollevare le saracinesche dei propri negozi o dei propri stabilimenti e garantire posti di lavoro, stipendi e futuro alle proprie famiglie e a quelle dei loro dipendenti, tra mille difficoltà economiche e burocratiche, affannati da una pressione fiscale ancora troppo alta, essi scopriranno che, anche grazie a quanto abbiamo fatto in quest'Aula, il loro vicino potrà lucrare sotto una finta etichetta sociale e potrà beneficiare di vantaggi fiscali e previdenziali, forse di incentivi economici, e probabilmente anche dell'impunità in caso di violazioni in tema di sicurezza o dei diritti dei lavoratori. Signora Presidente, questo sarà tutto molto sociale, ma non ci piace e per questo voteremo contro il disegno di Signora Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, il disegno di legge delega per la riforma del terzo settore giunge finalmente a conclusione, dopo una lunga discussione e un confronto articolato, che ne ha protratto per mesi e mesi l'esame. La proposta che adesso andremo a votare costituisce certamente una risposta organica - anche se non del tutto esaustiva - alle esigenze del volontariato e dell'associazionismo, che rappresentano da sempre realtà che rispondono a principi di solidarietà sociale e di equità, attraverso servizi e funzioni, che concorrono a formare un sistema di *welfare* diffuso e partecipato. Era particolarmente sentita l'esigenza di un quadro normativo organico e unitario, che fosse in grado di costituire un riferimento semplificato e al tempo stesso rafforzato e che restituisse capacità di sviluppo al mondo del volontariato, del *no profìt*, delle fondazioni e delle imprese sociali. Con il voto del Senato, si rinnova quindi, entro un quadro dinamico e flessibile, il rapporto indispensabile fra le istituzioni e quello che possiamo definire un ampio ed efficace insieme di reti di solidarietà. Sotto il profilo sostanziale, l'esercizio della delega si prefigura sempre più come una fase del procedimento legislativo. La definizione e l'approvazione dei principi di indirizzo sono sì un'espressione vincolante della rappresentanza e della volontà parlamentare, ma tuttavia rinviano all'adozione dei decreti attuativi la condizione decisiva affinché il processo di formazione della legge non si arresti. L'approvazione della legge delega è - per così dire - l'atto politico qualificato e propulsivo, sulla base del principio di autonomia del Parlamento che delibera e delega, ma la cui validità ed efficacia normativa dipendono dall'effettivo contenuto e dai tempi dei relativi decreti attuativi. La mia preoccupazione è che gli impegni assunti, certamente notevoli e numerosi - penso, ad esempio, all'annunciata revisione in materia tributaria, magari ad un vero e proprio codice

principi e indirizzi della delega abbiano la più efficace attuazione possibile. Il mio appello, dunque, è - e non potrebbe essere altrimenti - di procedere ad una rapida elaborazione e definizione dei decreti relativi agli indirizzi approvati con il voto sul disegno di legge delega, senza dover attendere il limite temporale dei dodici mesi previsto. Il settore attende, infatti, da anni segnali concreti di novità. Il Governo, sulla scorta anche dell'emendamento presentato dal relatore, sappia poi distinguere e riconoscere il vero volontariato e la sua validità sociale, da realtà che, in particolare nel volontariato organizzato che usufruisce di risorse pubbliche, appaiono estranee alle ragioni e al molo sociale del terzo settore. Vi sono tre ragioni costitutive della riforma del terzo settore che - a mio giudizio - devono essere in primo piano. La prima ragione è che una semplificazione del quadro normativo, entro una normativa nel contempo più cogente e omogenea, accresce opportunità e diritti; opportunità del mondo del volontariato e dell'associazionismo ad avere una legislazione alternativa ai vincoli esclusivamente burocratici che oggi rendono difficile, se non impossibile, la vita delle associazioni e delle organizzazioni che operano nel volontariato e nel *no profìt*. Si introducono così le basi per una crescita entro condizioni sostenibili del terzo settore; condizioni che rappresentano un rafforzamento dei diritti di cittadinanza, e dunque di partecipazione, a un sistema di *welfare* che, sia sotto il profilo economico che sul piano culturale, sia contraddistinto dall'obiettivo fondamentale di includere e non escludere i cittadini, secondo un approccio e un'offerta più mirati alla persona, quasi su misura e non standardizzati, e - come il disegno di legge ribadisce - con un'attenzione particolare alle persone e anche ai lavoratori più svantaggiati e bisognosi di tutela. È anche per queste ragioni che, nel mio impegno parlamentare, ho sempre ritenuto il terzo settore come una priorità: non soltanto come sistema integrato di servizi sociali e culturali, ma come possibilità di risposta, di accoglimento di istanze e aspettative che, altrimenti, avrebbero un ruolo ingiustamente marginale o, in ultima analisi, non riconosciuto nel nostro sistema economico e sociale. Penso al rapporto pubblico-privato, in favore di una regolazione più complessa dei soggetti sociali ed economici, che possa sostenere, nell'ambito delle risorse disponibili, una rete di tutele altrimenti negate. La seconda ragione è nell'impegno parlamentare che ho avuto su questi temi. Le nostre proposte, in parte presentate in occasione dell'esame della legge di stabilità o di altri provvedimenti attinenti del Governo, al di là delle motivazioni avverse relative alla sola copertura finanziaria, avevano esattamente l'obiettivo di ridurre vincoli; dare opportuna attenzione ai modelli flessibili e, per questa ragione, così ampiamente presenti sul territorio; valorizzare la ricerca e la programmazione delle compatibilità possibili per assicurare un quadro di prospettiva, e non esclusivamente contingente, alle forme di sostegno sociale ed economico garantite dal volontariato o dall'associazionismo. Purtroppo non ho ottenuto finora molta attenzione dal Governo, ma anzi posso dire che molte delle esigenze del settore *no profìt* sono state sottovalutate, probabilmente perché ritenute ingiustamente marginali. La terza ragione è che il modello di *governance* e di convivenza rappresentato dai territori di montagna - del Trentino nel mio caso è un esempio di quanto il terzo settore abbia e possa avere una storia e un ruolo strategico sotto il profilo economico, sociale e culturale. Il volontariato e l'associazionismo sono state le realtà che hanno garantito più opportunità di accesso all'economia e alla cultura, in ragione della diffusione capillare nel territorio, che è una risorsa del carattere distintivo del terzo settore e della sua unicità, come è la realtà del Trentino e dei suoi paesi di montagna. Non a caso il disegno di legge prevede anche la possibilità di promuovere la cultura del volontariato nelle scuole. Per questa ragione ho presentato in particolare due ordini del giorno che sono stati accolti, con qualche modifica, dal relatore e dal Governo e per questo li ringrazio. Il primo - e su questo il sottosegretario Bobba si è già attivato e lo ringrazio ha lo scopo di attuare una complessiva razionalizzazione delle modalità di richiesta della partecipazione al riparto del 5 per mille dell'IRPEF a carico di ONLUS, cooperative sociali, organizzazioni sportive dilettantistiche, organizzazioni non governative, enti del volontariato, organizzazioni di promozione sociale, e valutare, eventualmente, la possibilità di sanare

Il secondo ordine del giorno ha l'obiettivo di fornire un'interpretazione chiarificatrice dei collaboratori tecnici, comprendendo tra questi coloro che effettuano prestazioni di natura non professionale per l'espletamento dell'attività bandistica. Mi auguro che il Governo dia al più presto un'interpretazione, per non bloccare questo settore, che è vitale per la crescita culturale dei nostri territori, soprattutto dei più isolati. Ai medesimi criteri e obiettivi di crescita delle associazioni di volontariato, intese come ONLUS, erano ispirate le mie proposte di estendere l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro; di prevedere, al di sotto dei 30.000 euro, l'esonero dalla dichiarazione dei redditi per le associazioni dilettantistiche, in primo luogo per le *pro loco*; di stabilire l'esonero dal pagamento dei diritti di autore per le organizzazioni di volontariato e per le associazioni di promozione sociale che siano responsabili dell'organizzazione di iniziative a scopo puramente benefico; la possibilità di detrarre fiscalmente i costi per i corsi di formazione artistica a favore dei giovani allievi in campo musicale o coreutico. Si tratta di proposte che richiamano e ripropongono i contenuti di un disegno di legge presentato in questa legislatura a mia prima firma. Prendo atto dei vincoli derivanti dalle compatibilità finanziarie che oggi impediscono un loro accoglimento nel provvedimento di delega, ma ritengo sia importante che tali proposte siano riprese in altri provvedimenti del Governo. La disponibilità del sottosegretario Bobba a un confronto aperto nel corso dell'esame della delega, che ho apprezzato, così come del relatore Lepri, nel corso dello scrupoloso e attento lavoro in Commissione, ci fanno ben sperare. Dichiarando il voto favorevole del Gruppo Per le Autonomie-PSI-MAIE, mi auguro che finalmente il terzo settore, in tutte le sue articolazioni, possa ottenere l'attenzione che merita. Questo è un mondo che troppo spesso si è sentito dimenticato e che finalmente deve trovare la giusta dignità, per le persone che riesce a coinvolgere, per i numerosi esempi di responsabilità e sensibilità che fornisce, ogni giorno e dappertutto, soprattutto ai giovani, per aiutarli a diventare cittadini attivi, ma anche per la professionalità che ha raggiunto, per le economie che ha saputo realizzare e per i posti di lavoro che ha creato. Presidente, arriviamo dopo un lungo *iter*, anche in Commissione, al voto finale sul disegno di legge delega di riforma del terzo settore, che - lo dico con chiarezza - si aspettava da molto tempo. infatti, chiaro a tutti come vi fosse un'assoluta necessità di dar vita a una nuova legislazione che riordinasse e armonizzasse le varie leggi e norme di settore che si erano stratificate nel tempo,

forse, anche nella discussione di questi giorni, non sono stati tenuti ben presenti. Stiamo parlando di quasi 300.000 associazioni, cooperative, enti di volontariato, ONLUS moltissimi dipendenti. Stiamo parlando, tra l'altro, di 600.000 dipendenti diretti, 300.000 esterni: un mondo che ha dato, in tutti questi anni, un contributo enorme anche allo sviluppo del nostro Paese, uno strumento fondamentale - lo voglio qui ricordare - di grande inclusione sociale.

ad approcciarsi per indirizzare questo mondo non tanto nell'integrazione del *welfare* quanto addirittura in un meccanismo di vera e propria sostituzione (lo vedremo sulla questione della fondazione).

visto il tempo trascorso da quando è stato presentato ad oggi - sono passati circa due anni - un lavoro così importante di riordino e riforma si poteva assolutamente affrontare senza la delega. Lo dico perché, purtroppo, non possiamo dimenticare

noi continueremo a seguire questo provvedimento in modo molto puntuale e preciso, proprio e soprattutto nella parte che riguarderà gli schemi dei decreti legislativi.

Questo è per noi un elemento di preoccupazione enorme, perché nei tre anni trascorsi abbiamo visto, purtroppo, una dilatazione estrema dell'uso della delega per cui qui si legifera o con decreti-legge seguiti dalla fiducia o con il sistema della delega.

assolutamente recuperato. Voglio anche spendere qualche parola - ho sentito argomentazioni che non condivido affatto - sull'articolo 8, su cui noi - per esempio - abbiamo espresso un voto a favore. Si è presentato il ripristino del servizio civile universale addirittura come un *escamotage* per poter avere la preferenza nei concorsi pubblici,

del nostro Stato e cosa significa far riferimento ai valori costituzionali. Questo lo volevo dire con molta chiarezza, perché,

atti. Disconoscere quello che è stato e quello che potrà essere il valore del servizio civile universale credo sia un errore, proprio per i nostri valori costituzionali.

escludere l'articolo 6 da questo provvedimento, perché non si fa un favore alle imprese sociali vere se si continua a permettere che anche nell'impresa sociale

L'ultima questione riguarda l'introduzione, da parte del Governo, di un aspetto che non c'entrava assolutamente nulla. Come ha detto la mia collega Petraglia, la fondazione per finalità filantropiche si poteva fare da un'altra parte; penso e continuo a ritenere che essa non dovesse trovare cittadinanza all'interno di questo provvedimento. Ci sono due pericoli. Innanzitutto, come vedremo, essa svolgerà un ruolo negativo dal punto di vista del *dumping*, per quanto riguarda proprio il fatto di drenare tutte le risorse a disposizione delle associazioni, in un momento difficile. L'abbiamo detto tutti: perché bisognava intervenire per rilanciare il terzo settore? Perché siamo in una situazione difficile dal punto di vista sociale ed economico e quindi non bisognava fare concorrenza sleale alle piccole e medie associazioni che vivono del contributo dei privati. L'altro pericolo che è tutto insito, per quanto il testo sia stato modificato rispetto a quello che era stato presentato in Commissione - è che questa fondazione addirittura prende le risorse, le redistribuisce per le proprie finalità e, tra l'altro, rischia ancora una volta di essere un elemento sostitutivo del *welfare*; esattamente il contrario di quello che, come abbiamo detto fin dall'inizio, doveva essere lo scopo del riordino e di una riforma seria del terzo settore.

abbia creato ulteriori problemi, alcuni dei quali erano già presenti nell'impostazione del disegno di legge quindi tentato di dare il nostro contributo; abbiamo ottenuto certamente dei risultati di miglioramento rispetto al testo che proveniva dalla Camera; rimangono però a nostro avviso

Signora Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, signor sottosegretario Bobba quello di cui abbiamo discusso e che approveremo oggi è un provvedimento importante che in Italia si attende da molto tempo.

l'associazionismo *no profit*, le fondazioni e le imprese sociali. Come sappiamo, il concetto di terzo settore deriva dalla considerazione dell'esistenza, nel sistema economico e sociale, di un primo settore (ovvero lo Stato) e di un secondo settore (ovvero il mercato). Esso inquadra l'insieme di attività produttive che non rientrano né nella sfera dell'impresa capitalistica tradizionale, poiché non ricercano un profitto, né in quella delle pubbliche amministrazioni; ovvero abbraccia tutte quelle realtà che all'interno del nostro sistema socio-economico si collocano a metà tra Stato e mercato. Detto più semplicemente, gli attori del terzo settore operano nell'assistenza sociale, nella sanità, nella cultura, nello sport, nella cooperazione internazionale e nel volontariato; esse sono realtà che hanno natura giuridica privata (pensiamo alle cooperative sociali, alle associazioni di promozione sociale, alle organizzazioni di volontariato e non governative, alle ONLUS) che promuovono le loro attività senza fine di lucro. Il terzo settore ha registrato negli anni una costante crescita, nonostante l'ultima crisi economica europea che ben conosciamo. L'ISTAT ha censito oltre 300.000 organizzazioni *no profit*: una rete socio-economica che impegna 681.000 addetti, 271.000 lavoratori esterni e 6.000 lavoratori temporanei, mentre i volontari sono oltre 4,8 Date queste cifre, ci troviamo quindi di fronte ad una realtà importante e virtuosa del nostro Paese. Un settore che rappresenta addirittura il primo erogatore dei servizi per i cittadini; basti pensare che il mondo del *no profit* rappresenta il 4 per Nel 2014 si è svolta una consultazione pubblica sulle direttrici della riforma indetta dal Governo, e il disegno di legge successivamente presentato (sempre dal Governo) ha tenuto conto dei risultati ottenuti attraverso la partecipazione di tutti i soggetti interessati. L'anno scorso, il 9 aprile, la Camera ha approvato un testo migliorato che è arrivato all'esame della Commissione affari costituzionali del Senato, che, con ulteriori emendamenti, ha rafforzato l'obiettivo di fondo della riforma, ovvero creare un quadro normativo che favorisca la partecipazione attiva e responsabile delle persone, come singoli o in formazioni sociali di aggregazione, per tradurre i margini di crescita e occupazione dell'economia sociale in opportunità concrete per il settore e per il Paese in generale. Il riordino e la razionalizzazione degli incentivi economici e degli altri strumenti di sostegno mirano anche ad uniformare e coordinare una normativa di settore che nel tempo si è stratificata in modi anche disomogenei, per formare un quadro non più rispondente alle esigenze di regolazione e governo di queste fondamentali esperienze sociali. Diverse per struttura organizzativa (associazioni riconosciute e non riconosciute, fondazioni, comitati, cooperative sociali, associazioni ed enti di promozione sociale, organizzazioni di volontariato, organizzazioni non governative, società di mutuo soccorso, imprese sociali e ONLUS), le realtà del terzo settore hanno in comune alcune caratteristiche fondamentali, tra le quali, come già sottolineato, l'assenza di scopo di lucro, il che si traduce nell'obbligo di reinvestire gli utili nelle attività istituzionali, e la natura giuridica privata. Entrando brevemente nel merito del disegno di legge sottolineo i punti più qualificanti che il Gruppo parlamentare di Area Popolare ha sostenuto. Innanzitutto la revisione normativa che dovrà riguardare il terzo settore con la redazione di un apposito codice del terzo settore che preveda una disciplina unitaria; in modo condivisibile è previsto che le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche e le fondazioni bancarie siano escluse. Pertanto, con questo provvedimento si mira a riconoscere e garantire il più ampio esercizio del diritto di associazione e il valore delle formazioni sociali liberamente costituite, ove si svolge la personalità dei singoli, quale strumento di promozione e di attuazione dei principi di partecipazione democratica, solidarietà, sussidiarietà e pluralismo. Ma, onorevoli colleghi, non si può parlare di terzo settore senza avere ben presenti due concetti chiave che il disegno di legge valorizza: quello di solidarietà e quello di sussidiarietà. La solidarietà ha come suo significato principale una forma di impegno personale etico-sociale a favore degli altri. D'altra parte, siamo tutti consapevoli come la solidarietà possa esprimersi solo integrandosi con le politiche sociali del Paese in una convergenza trasparente ed efficace. Proprio per questo il Governo, riformando il terzo settore, dovrà individuare le attività di interesse generale che, svolte attraverso il più ampio accesso da parte degli interessati, presentino anche i requisiti per godere delle agevolazioni previste dalla normativa. Queste attività, individuate tenendo conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e differenziate in base al tipo di ente, sono gli elementi che, come detto, caratterizzano lo spirito e la finalità del provvedimento. Affinché il meccanismo di solidarietà sociale funzioni in modo virtuoso devono altresì essere stabiliti parametri e regole di funzionamento degli enti del terzo settore: questi dovranno essere organizzati e amministrati secondo principi di democrazia, eguaglianza, pari opportunità, partecipazione di associati e lavoratori, trasparenza, economicità gestionale e non potranno distribuire utili. Per quanto concerne la sussidiarietà, va nella giusta direzione la previsione secondo la quale deve essere valorizzato il coinvolgimento degli enti del terzo settore nella fase di programmazione territoriale dei servizi socio-assistenziali e di tutela dei beni culturali, con affidamento di servizi di interesse generale, valutando poi i risultati conseguiti. Un altro elemento caratterizzante il terzo settore è certamente il volontariato. Sul punto la riforma prevede una ricognizione e un riordino normativo che favorisca partecipazione, democraticità e gratuità delle attività di questi enti. Il volontariato viene inteso anche come promozione da parte dei giovani di iniziative solidaristiche, le cui competenze acquisite dovranno essere riconosciute in ambito scolastico e lavorativo. Ma, la riforma riguarda anche l'impresa sociale, la quale dovrà essere inquadrata come organizzazione privata che svolge attività d'impresa per finalità anch'esse civiche, solidaristiche e di utilità sociale, destinando i propri utili prioritariamente allo svolgimento delle attività statutarie e favorendo il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività ed auspichiamo che i decreti attuativi chiariscano in modo netto il suo oggetto, per evitare situazioni opache, anche raccogliendo sollecitazioni e perplessità evidenziate nel dibattito. Il disegno di legge, come già accennato, riforma anche il servizio civile, finalizzato alla difesa non armata della Patria e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, che rappresenterà, come ha affermato il presidente della Repubblica Mattarella, «un luogo concreto di protagonismo dei giovani (...) dove matura la loro piena cittadinanza, intesa come diritti e doveri, e dove possano crescere le loro opportunità». Si parla di opportunità di crescita, di conoscenza, di acquisizione di competenze per entrare nel mercato del lavoro. Ben 100.000 giovani ogni anno potranno accedervi e spetterà quindi allo Stato programmare ed organizzare, con il coinvolgimento delle Regioni, i piani specifici da parte di enti locali ed enti di terzo settore, i quali potranno attivare autonomamente progetti di servizio civile con risorse proprie. Un'ulteriore misura di razionalizzazione riguarda la registrazione di tali enti: sarà istituito un registro unico del terzo settore, al quale tutti gli enti che si avvalgano «prevalentemente o stabilmente» di fondi pubblici e privati, raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni e fondi europei dovranno, dovranno obbligatoriamente iscriversi. Ma la più forte e sentita considerazione che ci induce a votare favorevolmente questo provvedimento riguarda la cosiddetta questione sociale, che viene affrontata in questo disegno di legge. Viviamo un'epoca nella quale cresce il numero dei poveri e dei disoccupati soprattutto giovani, e nello stesso tempo, le istituzioni pubbliche fanno sempre più fatica a garantire prestazioni sociali di accettabile livello a tutti i cittadini. Oggi non si può dire che lo Stato, come previsto dalla Costituzione, faccia tutto il suo dovere per promuovere le condizioni sociali ed economiche e le condizioni amministrative ed istituzionali che rendono effettivo il diritto al lavoro. Proprio la questione sociale deve pertanto rimanere al centro dell'attenzione del dibattito politico, per l'importanza dei problemi che riassume, che affronta e che in molti casi prova a risolvere. prova a risolvere. Signora Presidente, con questa legge si mettono in moto le risorse migliori del Paese, le sue migliori energie, quella disponibilità a partecipare ad iniziative che contribuiscono al bene comune. L'essere umano è fatto per il dono, ma si devono favorire le condizioni perché si realizzi. Questa è la legge che vuole valorizzare e responsabilizzare la parte migliore della nostra Italia, che ogni giorno lavora gratuitamente e spontaneamente nelle nostre comunità, per portare aiuto ai bisognosi, a quelli che non hanno una casa, che sono privi di generi alimentari, agli anziani abbandonati, ai malati cronici senza assistenza domiciliare, e che per prima accorre quando si verificano calamità naturali. L'obiettivo finale è realizzare un'offerta integrata di interventi e servizi al fine di garantire il livello essenziale delle prestazioni. Un aiuto adeguato e mirato può mettere tante persone in condizione di uscire dallo stato di emergenza. Il terzo settore non è soltanto un impegno professionale, ma costituisce anzitutto una forma di missione e vocazione personale che si affianca alle attività lavorative ed extralavorative e agli impegni di vita e di famiglia, rappresentando veramente un servizio concreto per la comunità. Signora Presidente, per quanto detto finora, concludo dichiarando il voto favorevole del Gruppo Area Popolare

perché le firme apparenti sono quelle del Presidente del Consiglio dei ministri e del ministro Poletti, ma è evidente che non è stata fatta da loro (o, almeno, non solo da loro). Molti tra esponenti del Governo e colleghi di quest'Assemblea hanno legami e interessi con questo mondo ricco e diversificato. Ci sono però altri soggetti dietro le quinte: forse quel Vincenzo Manes, super consulente di Matteo Renzi, nonché finanziatore con 62.000 euro della sua Fondazione Open. stessa persona che parla di «una nuova IRI del sociale (...)», ossia «un grande fondo in cui confluiranno denaro pubblico, soldi privati e contributi di enti e fondazioni». Fondazioni che non si sa mai dove sono, cosa sono e chi sono. Guarda caso, durante l'*iter* di esame del provvedimento il Governo ha presentato un emendamento che va esattamente in questa direzione, apprestandosi di fatto ad appaltare la fondazione delle fondazioni nel terzo settore - mi riferisco a quella che hanno voluto chiamare Fondazione Italia sociale - al recinto dorato della Leopolda. Cosa proponevamo noi? Semplice: sostituire l'istituzione di questa fondazione con la reintroduzione dell'Agenzia per il terzo settore, cancellata dal Governo Monti. La fondazione pubblico-privata che vuole introdurre il Governo sarebbe invece l'ennesima mangiatoia e centro di potere in cui piazzare uomini vicini a Renzi e dalla quale gestire i flussi di finanziamenti, senza bandi o concorsi, nei confronti di progetti del terzo settore.

così - vanno rilevati anche alcuni aspetti positivi, come il nuovo codice del terzo settore, il registro unico degli enti del terzo settore, e i numerosi miglioramenti, come per esempio la previsione di regimi sanzionatori di cui non si parlava compiutamente. Ma, come fate da tre anni a questa parte, prima con Berlusconi e oggi con Verdini, le due cose buone che riuscite a mettere in fila servono solo ad andare in televisione a prendere in giro gli italiani dicendo che sicuramente si poteva fare meglio, ma che qualcosina avete fatto; come se ci fosse un'entità astratta che vi trattiene dal fare bene una cosa giusta dall'inizio alla fine. non c'è una entità astratta, ma un obiettivo concreto: veicolare interessi clientelari e di controllo del consenso attraverso mezzi normativi improntati esteriormente a finalità filantropiche. *(Applausi del senatore È stato così per quell'obbrobrio di riforma elettorale che avete prodotto: con il pretesto fasullo di ridurre i costi (che non avete ridotto), avete consegnato la democrazia ai potentati partitocratici. È stato così per la "cattiva scuola" e per la "deforma" del mercato del lavoro. Predicate male e razzolate malissimo. Sul disegno di legge in esame votiamo contro per metodo, perché non se ne può più di deleghe al Governo che ha espropriato il Parlamento e ridotto la Repubblica parlamentare ad un parcheggio riservato ai clienti. Si tratta di deleghe fumose, ambigue, su cui finisce addirittura una norma bella e finita, come quella che che istituisce quella fondazione di secondo livello che nemmeno nella maggioranza - vivaddio! - è riuscita a risultare digeribile. L'Agenzia per il terzo settore che noi proponevamo sarebbe dovuta essere un organismo indipendente, costituito con lo scopo di coordinare le diverse realtà del terzo settore, fare da raccordo con gli enti locali, vigilare sui flussi finanziari; ma nello stesso tempo doveva essere sottratta alla cannibalizzazione della politica. La spina dorsale del terzo settore è etica, non finanziaria; è improntata a pluralità, sussidiarietà, vicinanza al territorio (anzi ai territori), non basata sulla spinta aggregativa in *holding* finanziate da privati che apre poi a speculazioni lucrative sulla gestione dei diritti civili e sociali. lo avete fatto includendo il fine di lucro, la remunerazione del capitale d'investimento, aprendo il terzo settore alla finanza, senza limiti al conflitto d'interessi, alla presenza negli organi di controllo delle cooperative

Non è solo una questione estetica: questa delega in mano al Governo rischia di peggiorare l'economia sociale del Paese: tante piccole realtà verranno stritolate a causa della posizione dominante garantita a pochi soggetti vicini al Governo. questi stessi saranno limitati nella loro indipendenza attraverso la discrezionalità nel dirigere gli investimenti e i finanziamenti. Con il disegno di legge in esame volevate addirittura cooptare i centri servizio volontariato ad una funzione spuria a vantaggio degli operatori economici del mercato. Del resto, non si escludono esplicitamente dal terzo settore - come chiedeva il Movimento 5 Stelle - le fondazioni politiche, cioè quella terra di mezzo in cui i soldi

anzi, molti di voi ne sono addirittura a capo, come nel caso di Altero Matteoli con la Fondazione della libertà per il bene comune, di Gaetano Quagliariello con la Fondazione Magna Carta, di Maurizio Gasparri con la Fondazione Italia protagonista, fino ad arrivare a Roberto Formigoni, cui fa capo la Fondazione Europa e civiltà, che si dichiara solo lombarda e dunque è sottratta al controllo statale.

è lievitato in poco tempo passando dai 20.000 euro iniziali agli oltre 2,8 milioni di euro. Se il Presidente del Consiglio fosse altrettanto interessato al Paese quanto lo è alla sua fondazione,

e privatistica, come è stato sancito con l'articolo che istituisce l'impresa sociale e include in essa anche le finalità di lucro e redistribuzione degli utili, con l'avallo del sistema politico e la circolazione di denaro in doppia direzione, in partita di giro, nei rapporti che conosciamo. Signora Presidente, noi non crediamo in questa visione di società che hanno Matteo Renzi e i suoi amici. Crediamo in una comunità improntata sulla partecipazione, sulla meritocrazia, sulla trasparenza, sulla libertà; libertà anche dal malaffare però, dalle clientele, dalle *lobby*, dalla criminalità organizzata e dai venditori di riforme "un tanto al chilo". Avevamo ben chiaro cosa si doveva premiare e cosa si doveva scongiurare. Avevamo l'occasione di dire al Paese che degenerazioni come quelle viste con Mafia Capitale non sarebbero più capitate, perché questi strumenti normativi avrebbero impedito di dubitare di un settore virtuoso per colpa di poche mele marce. Si è persa un'occasione e, signora Presidente, in politica l'omissione è colpa.

oggi abbiamo dinanzi a noi un disegno di legge delega al Governo sul terzo settore, scritto e modificato dal Governo stesso. A questo punto mi chiedo come mai non sia stato scelto lo strumento del decreto-legge, magari da blindare con una questione di fiducia. è anche peggio, perché l'Assemblea decide scientemente di ratificare una delega talmente vasta e generica, più simile ad una raccomandazione che ad un provvedimento vincolante. Quindi il Senato legifera per non legiferare: un vero paradosso legislativo. Siamo chiamati a rinunciare totalmente alla nostra funzione principale a favore di un Esecutivo che più volte ha dimostrato la sua incapacità nell'uso delle deleghe; una spoliazione di potere

Ma tornando al cuore del provvedimento, esso tratta del terzo settore: un mondo vario, multiforme, situato in posizione intermedia tra pubblico e privato di cui rappresenta il naturale collante, totalmente differente dal mondo di mezzo passato all'orrore delle cronache. Proprio in virtù di questa sua multiformità, si presentava non solo necessario, ma fondamentale un intervento regolatorio che semplificasse il panorama del *no profit*, che facesse maggiore chiarezza sul tema, soprattutto alla luce degli sviluppi penali che sempre più investono il mondo del *no profit,* e definisse limiti e confini specifici all'opera dei soggetti che costituiscono tale comparto. L'istituzione di un testo unico contenente tutte le norme del terzo settore, previsto dal provvedimento in esame è la giusta risposta a questa necessità ma, purtroppo, è anche l'unica nota positiva della delega, che per il resto è il solito pasticcio cui ci ha abituati un Esecutivo bravo nei titoli ed inconcludente nella sostanza. quelli che abbiamo imparato negli ultimi due anni, come quando questo Esecutivo ha definito «riforma» un provvedimento, che nasconde solo un riordinamento legislativo il cui reale beneficiario ed esclusivamente Palazzo Chigi: basti pensare alla riforma costituzionale, a quella della scuola e - non ultima - alla riforma del sistema bancario. La motivazione di tale interesse ce la offrono i numeri del terzo settore: parliamo di un giro d'affari pari a 64 miliardi di euro, in costante aumento negli ultimi anni, di un contributo lavorativo di 4,7 milioni di volontari, 681.000 dipendenti, 270.000 lavoratori esterni e 5.000 lavoratori temporanei. Nel tessuto produttivo italiano il *no profit* occupa pertanto una posizione significativa, con il 6,4 per cento delle unità economiche attive. Si capisce bene, quindi, il ruolo sostitutivo che il terzo settore ha rispetto alla erogazione dei servizi di *welfare*, laddove lo Stato, le Regioni e i Comuni continuano a latitare e a diminuire i propri servizi sociali a causa dei continui tagli lineari operati dalle più recenti leggi di finanza pubblica. Questo disegno di legge, come detto, avrebbe dovuto favorire le buone pratiche e contrastare gli illeciti; invece rappresenta solo un intervento utile al Governo per fare cassa e aumentare le proprie competenze e il potere su questo settore, aumentando la confusione, con la creazione di un modello di impresa sociale ibrido, che di sociale rischia di avere ben poco. Mi riferisco, in particolare, a quanto contenuto nell'articolo 6, che prevede che l'impresa sociale destini i propri utili prevalentemente al raggiungimento di obiettivi sociali. Ebbene, con la scelta dell'avverbio «prevalentemente» si crea una dicotomia per cui imprese che, avendo nel proprio oggetto sociale la creazione di un impatto materiale positivo sulla società erano vincolate a perseguire tale scopo, potrebbero d'ora innanzi esercitare legalmente un'attività di impresa capitalistica, pur continuando ad usufruire di finanziamenti pubblici. Si rischia di avallare con legge dello Stato una concorrenza sleale tra diverse tipologie di impresa del Paese. Ad aggravare questa situazione vi è l'articolo 7, che attribuisce le funzioni di controllo e monitoraggio del settore al Ministero del lavoro e delle politiche sociali mediante la promozione di forme di autocontrollo degli enti del settore: quindi creiamo una sorta di uroboro, per cui il controllato garantisce il suo stesso operato. Si tratta di una lacuna o di una disattenzione? No, si tratta di una scelta consapevole del Governo per aggirare ogni forma di controllo effettivo: prova ne è il reiterato rifiuto di modificare tale sistema includendo la collaborazione dell'Agenzia delle entrate o del *jolly* governativo, Sono queste le decisioni che rivelano come sia evidente che l'Esecutivo preferisce un settore dai confini indeterminati e fumosi. L'indeterminatezza, tuttavia, non si riscontra nell'attribuzione alla Presidenza del Consiglio del coordinamento delle politiche di governo e delle azioni di promozione e di indirizzo delle attività delle associazioni e dei soggetti del terzo settore. un accentramento di potere che Forza Italia non condivide e che riteniamo favorisca solo un maggiore appesantimento della struttura dello Stato centrale a scapito della competenza regionale in materia, riconosciuta dalla stessa Costituzione, e del principio di sussidiarietà. un tentativo di far diventare il terzo settore un terreno di caccia del Governo, palesatosi con il folle emendamento, in cui si prevede la creazione, con fondi pubblici, della Fondazione Italia sociale, presentato prima in Commissione, ma ritirato a causa della forte resistenza delle opposizioni, per essere poi nuovamente riproposto in quest'Aula e approvato pochi minuti fa, con solo una manciata di voti. una fondazione pubblico-privata, una nuova IRI del terzo settore, che riproduce fedelmente lo stile di Palazzo Chigi e della sinistra, abituata a creare carrozzoni di di carattere clientelare per consentire ai *Premier* di rastrellare finanziamenti per gestirli a proprio piacimento, senza bandi o concorsi, finanziando solo i soggetti di proprio interesse: l'ennesimo poltronificio statale, un po' come il futuro Senato. Ancora una volta, questo Governo ha dato conferma di come l'utilizzo del potere sia esclusivamente indirizzato al perseguimento dei propri scopi e non a favorire la reale ripresa del nostro Paese ed è per questo motivo e per le criticità esposte in precedenza che annuncio il voto contrario di Forza Italia. *(PD)*. Signor Presidente, senatrici e senatori, il dibattito svolto in quest'Aula, ma prima di questo anche quello svolto nell'Aula della Camera, ha dimostrato una ricchezza di esperienze che costituisce un solido vissuto, condiviso tra molti di noi. Il terzo settore ha trovato in questi anni spazi per uno sviluppo quasi tumultuoso, che ha mostrato tante potenzialità con esperienze di crescita e consolidamento, ma ha evidenziato anche la fragilità di esperienze piccole e frammentate. Il tempo dedicato al lavoro di confronto e di ascolto che è stato fatto in occasione di questa delega ci ha fatto capire quanto questo settore aspettasse questo provvedimento, ma anche quanto questo provvedimento fosse in qualche modo visto con preoccupazione. Si tratta di un mosaico che restituisce una vasta complessità, certo, ma restituisce pure la consapevolezza che occorre esercitare oggi la responsabilità per dare risposte che adeguino gli strumenti legislativi su alcuni aspetti, ne chiariscano altri e che soprattutto aprano nuove opportunità. Il volontariato vive di motivazioni forti che non possono trovare nel contesto legislativo elementi di preoccupazione, e la delega crea quel quadro che mancava per dare fiducia, pur rimandando alle varie leggi di settore, che vengono comunque riconosciute valide nella loro specificità e che comporranno parti del codice del terzo settore. Ma è proprio in questa sorta di dualismo fatto di miglioramento degli assetti attuali e di predisposizione a cogliere nuove possibilità che la delega si muove, perché ogni complessità porta con sé problemi e opportunità. solo ad adeguare un sistema di norme ad un mondo come quello del volontariato sarebbe sicuramente riduttivo per un mondo che, seguendo la gratuità, si evolve velocemente e non può che aprire nuove strade. Muovendomi su questa falsariga sottolineo alcuni aspetti di complessità, a partire dalle storie differenti che si sono sviluppate sul territorio nazionale. Il più volte richiamato articolo 118 della Costituzione è stato declinato nei diversi modi in cui le singole Regioni hanno coordinato l'attuazione della sussidiarietà. Pure i singoli modelli sociali e culturali che costituiscono la ricchezza del nostro Paese, hanno determinato differenze importanti tra i vari territori nell'organizzazione del terzo settore. Infine, gli spazi di integrazione che si sono sviluppati tra enti locali, terzo settore e tessuto imprenditoriale, nelle varie parti d'Italia hanno dato vita a contesti diversi. Per esempio, tanta cooperazione sociale è la naturale evoluzione del volontariato che sa affrontare le sfide della qualità, degli accreditamenti, della professionalità, contribuendo a dare risposte appropriate in un quadro di sussidiarietà dove l'ente pubblico non si disfa dei servizi perché poco capace, ma al contrario, proprio perché ente pubblico capace ed efficiente, sa organizzare la gestione integrata dei servizi. Sempre sul fronte dell'imprenditoria sociale la delega scioglie alcuni vincoli della disciplina attuale (il decreto legislativo n. 155 del 2006) che potranno permettere ad un maggior numero di organizzazioni di acquisire la qualifica. Al contempo gli strumenti innovativi per le imprese sociali dovranno essere presto agibili e di semplice utilizzo per essere messi in campo, a fronte di una serie di bisogni emergenti: ad esempio, le nuove povertà che possono essere affrontate con percorsi mirati di reinserimento lavorativo che attivino le persone e le sfide demografiche, l'invecchiamento della popolazione e la richiesta crescente di servizi residenziali e domiciliari. L'imprenditoria sociale e i settori in cui opera è già oggi una fonte di occupazione giovanile. Può diventare una miniera di posti di lavoro per i giovani, ad esempio, nel settore del turismo sociale e dell'agricoltura sociale, sopratutto nel Mezzogiorno. Allo stesso modo le diverse storie regionali dei centri di servizio per il volontariato rapportate al tessuto associativo, con la delega si aprono ad un futuro capace di sostenere l'articolazione attuale e ad accogliere le novità che stanno già nascendo. Un altro elemento di complessità è la gamma dimensionale caratterizzante il nostro terzo settore, fatto spesso di piccole entità capaci di capillarità ma non sempre di organicità, con deboli reti di secondo livello che ora vengono riconosciute e valorizzate attraverso il Consiglio nazionale del terzo settore. La disomogeneità della forma organizzativa e societaria degli enti di terzo settore a volte crea instabilità. Con la delega vengono chiarite bene le differenze tra le diverse formule organizzative del terzo settore, obiettivo centrale che il Governo aveva sottolineato. Con i decreti delegati si dovranno riscrivere le regole che si applicano in un'ottica di chiarezza e semplicità e dovranno mettere in campo strumenti innovativi adeguati a fornire risposte ai bisogni emergenti cui oggi complessivamente il terzo settore fa fronte. I controlli dovranno essere sostanziali e non formali o macchinosi. Da questo punto di vista è importante che i decreti definiscano a monte le regole in modo chiaro e semplice, in particolare sulla disciplina fiscale. Sotto questo profilo è centrale e decisivo il nuovo codice degli appalti su cui il Parlamento sta lavorando. Un pensiero specifico va ai giovani. Una riforma del terzo settore che non sapesse fare spazio ai giovani sarebbe un fallimento, anche pensando a quello che è sotto i nostri occhi e cioè il progressivo aumento dell'età media della popolazione, anche quella dei volontari. Pensare ai giovani significa immaginare che la gratuità di cui sono capaci deve potere scrivere nuove storie, percorrere nuove strade, occuparsi di nuovi bisogni, arricchire di sensibilità le nostre comunità, trasformare lo slancio in competenze. Un esempio su tutti che l'attualità ci propone come un *link* chiaro ed evidente è rappresentato dalla lotta allo spreco alimentare, con un progetto di legge da poco approvato alla Camera: un nuovo ambito di impegno di volontariato e non solo che incontra l'attenzione proprio dei giovani. Qui si innesta la riforma del servizio civile universale: è uno degli aspetti su cui il Governo ha puntato di più. Ora la riforma deve essere il volano per focalizzare le politiche giovanili su questo istituto che per l'attivazione dei NEET (giovani NEET *not in education, employment or training*) si è rivelato, in questi anni, uno strumento eccezionale.

Importante è anche l'inserimento volto a «garantire, negli appalti pubblici, condizioni economiche non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro adottati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative». la revisione totale del sistema dei centri servizio volontariato, a cui possono concorrere tutti gli enti del terzo settore, salvo le cooperative sociali e le imprese sociali, e il superamento del sistema degli osservatori nazionali per il volontariato e per l'associazionismo di promozione sociale, attraverso l'istituzione del Consiglio nazionale del terzo settore,

Cambia la qualificazione dell'impresa sociale e se ne chiarisce la collocazione all'interno del terzo settore, superando, opportunamente, la definizione *f)* della Camera, che individuava l'impresa sociale per l'obiettivo di «generare un impatto sociale positivo», collocando invece in modo appropriato le tematiche dell'impatto nell'articolo 7. Per i settori, ora è previsto che saranno individuati all'interno delle attività di interesse generale complessive per il terzo settore, che saranno definite nei decreti legislativi. Cambia la formulazione della distribuzione degli utili nelle imprese sociali con una formula più precisa e coerente prevista la ridefinizione delle categorie di lavoratori svantaggiati, tenendo conto delle nuove forme di esclusione sociale, anche con riferimento ai principi di pari opportunità e non discriminazione. inserito l'obbligo di bilancio *ex* codice civile per le imprese sociali. Laddove un ente del libro primo del codice civile assuma la qualifica di impresa sociale si sottopone agli stessi obblighi fondamentali di trasparenza contabile propri delle imprese. Avviandomi a concludere, aggiungo che è fondamentale che gli oneri burocratici che tutte le organizzazioni esistenti dovranno affrontare per far fronte alle novità della riforma siano semplificati al massimo e non siano onerosi per il terzo settore. Se affrontiamo il capitolo delle risorse messe in campo, è opportuno richiamare le principale scelte fatte dal Governo Renzi. Con la legge di stabilità 2015 abbiamo stabilizzato il 5 per mille con una dotazione di 500 milioni di euro ed abbiamo innalzato a 30.000 euro all'anno (rispetto ai precedenti 2.065 euro) l'importo massimo detraibile Un decreto MISE dell'anno scorso istituisce «un regime di aiuto volto a sostenere la nascita e la crescita delle imprese operanti, in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento degli interessi generali e delle finalità di utilità

euro. Con la legge di stabilità 2016 abbiamo già inserito le dotazioni per l'attuazione della riforma che approveremo tra poco: 140 milioni di euro per il 2016 che diventano 190 nel 2017 e nel 2018. Infine il fondo progetti per

con questo strumento non si cambia il segno della riforma, entrando a gamba tesa sul terzo settore e facendo concorrenza sleale rispetto ai soggetti che raccolgono risorse private. Si mette invece in campo uno strumento che cerca da una parte di recuperare risorse che oggi nessuno riesce a recuperare, per metterle da un'altra parte, a disposizione di progetti di ampie dimensioni. Per fare questo occorre un soggetto strutturato e credibile, che consenta a questa tipologia di donatori, che oggi nessuno riesce ad attivare, di rendersi parte attiva nel campo sociale. Questa Questa riforma interviene ad aggiungere un altro tassello al processo di modernizzazione che stiamo imprimendo al Paese. Se mi permettete di muovermi sul filo di un doppio senso, dico che la nostra società è vero che ha bisogno di adeguare le proprie istituzioni, è vero che deve diventare più competitiva nel suo tessuto produttivo, è vero che deve investire nella scuola, ma, come tutte le società che vogliono fare investimenti, deve essere capitalizzata. Ecco, con questa riforma facciamo un aumento di capitale sociale dell'Italia. Dichiaro pertanto il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico.

mi unisco ai ringraziamenti del relatore, a cominciare da lui stesso, dalla Presidente della Commissione e da tutti coloro che hanno operato. È stato un lavoro - come qualcuno dei senatori ha ricordato - che non è stato per nulla compresso.

nell'articolo 118 della Carta costituzionale riformata nel 2001, cioè quindici anni fa, secondo cui le istituzioni tutte, a cominciare dal Senato, «favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento

che ancora una volta la Sardegna è vittima di una piaga criminale ormai intollerabile, intollerabile, che colpisce con attentati vigliacchi i beni, le case e le persone che si dedicano all'amministrazione pubblica. una piaga che è stata una piaga che è stata alimentata in questi anni dall'aggressione sistematica, puntuale e sempre più feroce verso la politica che non fa distinzioni tra coloro che dedicano la propria esistenza all'interesse generale e coloro che, invece, approfittano della politica per ottenere illeciti arricchimenti. Tanti amministratori locali onesti, tanti sindaci di piccoli Comuni, tanti giovani consiglieri comunali, nelle terre del disagio e dello svantaggio, rischiano puntualmente la propria vita per dedicarsi all'interesse generale, per sostenere nei modi più utili possibili i diritti dei cittadini che amministrano. In questi giorni c'è una recrudescenza fortissima in Sardegna: sono state colpite amministrazioni locali prevalentemente dell'area del nuorese e delle zone interne della Sardegna. In questa legislatura, attraverso In questa legislatura, attraverso la Commissione ben diretta e governata dalla collega Lo Moro con grande impegno e con grande garbo, abbiamo affrontato il problema delle intimidazioni e degli attentati agli amministratori locali della Sardegna e di tutto il resto d'Italia, e abbiamo definito e approvato unanimemente in quest'Aula alcune proposte che sono state avanzate al Governo. Tali proposte sono contenute nella relazione conclusiva dei lavori di quella Commissione, ma sono ancora sostanzialmente

Queste proposte noi le riproponiamo al Governo e lo faremo con un'iniziativa congiunta di diversi parlamentari della Sardegna, per richiamare anche

concludersi con l'espressione di solidarietà mia e del mio Gruppo verso tutti gli amministratori locali della Sardegna, e non solo, che hanno subito intimidazioni e attentati in questi giorni. Signor Presidente, colleghi, in Sicilia accadono fatti inquietanti accadono fatti inquietanti che, senza un'attenta informazione, ma soprattutto senza il coraggio di quegli amministratori che alzano la testa e denunciano, resterebbero nascosti nei meandri della burocrazia. Accade che a Furnari, in provincia di Messina, un terreno di proprietà della Regione Siciliana, che nel 1991 era stato stimato per un valore di 300 milioni di vecchie lire, venticinque anni dopo, nel 2016, venga svenduto per meno di 4.000 euro. Accade che la fortunata acquirente sia imparentata con il responsabile del procedimento dell'ufficio del genio civile di Messina. Accade che il procedimento in questione risulti vistosamente viziato da plurime irregolarità e illegittimità denunciate per tempo. Accade, infine, che, a seguito della denuncia, del sindaco di Furnari, la storia è stata portata alle cronache da una nota trasmissione televisiva e soltanto allora il governatore siciliano Rosario Crocetta sembra essersi accorto della vicenda. Accade che lo stesso Crocetta abbia subito annunciato grandi azioni di verifica della regolarità delle procedure, ma accade anche che l'avvocatura dello Stato, in rappresentanza dell'amministrazione regionale da lui guidata, lo abbia smentito nei fatti giustificando la svendita dell'immobile. Quello di Furnari, colleghi, non è affatto un caso isolato. Anche nei Comuni di Porto Empedocle e Stromboli si registrano compravendite tra la Regione Siciliana e soggetti privati a seguito di pagamenti di somme irrisorie. Il legame di parentela tra i protagonisti della vicenda è quanto mai inquietante e non sorprende che il governatore Crocetta, ancora una volta con le spalle al muro, abbia scelto di nuovo il gioco delle tre carte. Ancora, Crocetta racconterà della mano destra che non sa quello che fa la sinistra, ma questa volta stiamo avvisando noi il Governo nazionale per tempo. Anche a Stromboli e Porto Empedocle la Regione ha svenduto a privati in cambio di somme risibili.

il grande inganno della commissione grandi rischi è ancora presente purtroppo nella mente degli aquilani, al punto che è si è svolta questo pomeriggio una manifestazione per ricordare quella buffonata mediatica con la quale il 30 marzo 2009 il *team* degli scienziati, sotto l'insipiente guida del comandante Bertolaso, rassicurò la popolazione sui rischi e pericoli di imminenti gravi scosse sismiche. Non si può assolutamente allarmare, ma non si può neppure rassicurare. Guido Bertolaso, vergognosamente tornato sulla scena politica di Roma con la sua candidatura a sindaco, fortemente voluta dal "berlusconiano" Berlusconi, è imputato nel processo grandi rischi *bis* e ha un'imputazione per reati di omicidio colposo plurimo e lesioni per quella telefonata che fece all'*ex* assessore regionale abruzzese alla protezione civile, nella quale preannunciava la famosa riunione del 30 marzo come un passaggio unicamente mediatico per rassicurare la popolazione da eventuali rischi di scosse sismiche. Passaggi mediatici che ha imparato anche il signor Renzi. La telefonata, secondo l'accusa, ebbe l'effetto di indurre gli scienziati partecipanti alla medesima riunione a sostenere che la necessità di evitare gli allarmismi e valutare con superficialità il reale rischio di quello che sarebbe accaduto era cosa necessaria. Il signor Bertolaso ha più volte annunciato nelle ultime settimane di non volere scappare dal processo, ma di ritenere doveroso sottoporsi al pieno giudizio del tribunale di L'Aquila. Allora, agli annunci finora non sono seguito i fatti visto che ancora non ha depositato alcun atto formale.

che va fatto presso la cancelleria del tribunale aquilano, come viene sbandierato in tutte le trasmissioni. La collega, all'epoca anche lei accanto ai politici del territorio, si faccia dunque portavoce di questa necessità. Per quanto tempo ancora Bertolaso ha intenzione di prendere in giro i cittadini romani?

se ci sono state anche delle *trastole* all'interno dei *software* che gestiscono le liste. **Mozioni,

e 4 decessi. Nel 2015, sempre in Toscana, i casi sono stati 38 e le morti 7. I casi di meningite non si arrestano. La Regione Toscana sta facendo il massimo e l'assessore Saccardi continua giustamente a rinnovare l'appello a vaccinarsi, ma occorrerebbe promuovere

e i centri vaccinali ampliando gli orari delle vaccinazioni e incrementando le risorse. Soprattutto, occorrerebbe che l'Istituto superiore di sanità

Presidente, siamo preoccupati perché solo qualche giorno fa all'assemblea annuale di Confcooperative veniva descritta un'Umbria in difficoltà, che non riesce ad agganciare la ripresa, ma soprattutto ci sono dati statistici che testimoniano di un declino marcato: -8 per cento rispetto al PIL delle altre Regioni italiane. È proprio di queste ore la notizia che il collegamento Roma-Perugia gestito da Etihad, ovvero da Alitalia, sarà soppresso e sostanzialmente portato a zero. Questo ci preoccupa molto perché una Regione operosa verrà completamente tagliata fuori e dimenticata dal sistema dei collegamenti nazionali.

viario, viene da chiedersi se siamo in Italia o nel Terzo mondo. Non ci sono politiche in atto da parte della Regione e non si vedono politiche da parte dello Stato e del Governo. Su queste materie occorre essere chiari: o si fanno collegamenti oppure si resta tagliati fuori e il PIL non può che precipitare. Vogliamo delle certezze; vogliamo chiarezza da parte del Ministro.

rispetto alle tante parole di solidarietà che vengono spese in questo momento da parte di tutto l'apparato politico, a cominciare dal Presidente della Repubblica, dal Presidente della Regione Sardegna, dal Presidente del Consiglio regionale,